e non per la prima volta - per quanto riguarda l'obbligo di attrezzare gli impianti sportivi con defibrillatori semiautomatici,

e quali azioni si pensa di intraprendere per quanto riguarda questa responsabilità per i casi critici appena illustrati.

Signora Presidente, ringrazio i senatori per aver sollevato ancora una volta una tematica, per quanto riguarda il Ministro della salute, di indubbia rilevanza e, per le ragioni di tempistica che sono state descritte, anche di grande attualità, che mi consente di chiarire - spero con un'unica risposta, attesa l'analogia della tematica in esame la complessità della materia, in considerazione, soprattutto, del susseguirsi anche di interventi normativi e regolamentari, che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni. In via preliminare, parlare di defibrillatori, come è noto, equivale a riconoscere la valenza degli stessi in termini di sicurezza negli impianti sportivi. Questa normativa è nata dopo dopo eventi noti alla cronaca sportiva del nostro Paese, per molti aspetti drammatici, che quindi hanno determinato anche un effetto di iniziativa normativa assolutamente importante, non soltanto per la sicurezza degli impianti, ma anche per una specifica formazione degli operatori e per un'attività sempre più puntuale in termini di informazione sia degli atleti sia anche del pubblico.

dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito a sua volta dalla legge n. 98 del 2013, ha previsto specificamente che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici o di eventuali altri dispositivi salvavita. Per attuare la norma è stato adottato il decreto ministeriale del 24 aprile 2013 recante disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche si devono dotare di defibrillatori, seguendo le modalità dell'allegato E del decreto, con una tempistica notoriamente differente:

il termine è stato portato da trenta a trentasei mesi. Pertanto, come è stato segnalato, il termine per dotarsi dei defibrillatori scade in data 20 luglio 2016.

di formazione degli operatori, obbligatorie per l'utilizzo di questi strumenti, del settore sportivo dilettantistico che erano state già avviate, ma non concluse. Ritornando alle linee guida di cui all'allegato E del decreto, ricordo che le stesse stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.

ha già stabilito da anni i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori esterni quali dispositivi medici da utilizzare sia in strutture sanitarie, che in qualunque altro tipo di di strutture mobili, stabili o temporanee. Questo accordo del marzo 2011 regola ovviamente anche questa ulteriore attività, che è successiva. Per quanto riguarda l'ultima domanda posta nell'interrogazione della senatrice Idem, anche in queste ore

parzialmente soddisfatta della risposta perché il quadro normativo è molto chiaro e si è trattato di una risposta a emergenze verificatesi in passato. La risposta legislativa è assolutamente giusta per quanto riguarda sia la certificazione

adempiente rispetto alla legge. Mi spiego con parole molto semplici. Pensiamo a un ciclista che esercita il suo sport sulla strada, facendo tanti chilometri, a un canottiere e a un canoista che si trovano fuori dell'impianto acquatico o a un atleta che fa la maratona e si allontana dall'impianto sportivo. Qualcuno

perché nella maggior parte dei casi i presidenti delle associazioni sportive sono dei volontari che garantiscono con il proprio patrimonio personale.

in alcuni casi ha una conseguenza poco auspicabile. Le persone si ritirano, non si assumono più le proprie responsabilità e il tessuto della pratica sportiva rischia di assottigliarsi.

Sono contento e soddisfatto della sua sensibilità, però egli non ha risposto a parte dei quesiti che ho posto nell'interrogazione, soprattutto a quelli che che mi interessano di più. Sgombro subito il campo da ogni intenzione che non sia quella giusta e dico che la Provincia autonoma di Trento ha già attivato una legge che finanzia fino al 95 per cento della spesa per l'acquisto di defibrillatori. Nel nostro pur piccolo territorio, sono già più di 250 i defibrillatori acquistati e si pensa addirittura di mettere i defibrillatori in ogni quartiere della città di Trento. I defibrillatori infatti non interessano solo gli sportivi, perché una crisi cardiaca può capitare anche ad un cittadino che cammina per strada. Questa emergenza è assolutamente avvertita e tutto il volontariato che opera nel campo della salute e dell'emergenza già da anni è attivo. Quindi sgombriamo il campo da questo ragionamento.

sono persone che gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo, sono genitori che portano in giro i ragazzi, che seguono l'attività agonistica o sportivo‑dilettantistica a titolo gratuito

che gestisce contemporaneamente sei strutture sportive (parlo di calcio, naturalmente). Finita la scuola, i bambini vanno a giocare; ci sono sei squadre che contemporaneamente giocano in sei strutture. Va bene finché ci sono le partite, questo è garantito; ma proviamo a pensare agli allenamenti, proviamo a pensare a quando cinque o sei ragazzi si mettono a correre in un campo. Come fa una società a garantire la presenza di un addetto specializzato che si assuma la responsabilità, per tre o quattro ragazzi che si mettono a correre? correre? Qual è pericolo di questa norma? Che le strutture rimangano chiuse, perché nessuno si prende la responsabilità di tenerle aperte, e che alla fine andiamo a demotivare il volontariato sportivo, ma soprattutto la pratica dello sport.

del defibrillatore e dell'addetto è dovuta, riconosciuta e sacrosanta. Ma, nel momento in cui stiamo parlando di microallenamenti o di piccoli incontri sportivi fatti la sera dopo cena con alcuni amici, amici, rendere necessaria la presenza dell'addetto è un problema ed è soprattutto un problema renderlo responsabile. Quindi incentiviamolo e facciamo in modo che ci sia; ma obbligare la società a trovare, ogni volta che qualcuno entra in un campetto, chi si assume la responsabilità dell'uso corretto del defibrillatore per noi è un problema e significa creare, nel tessuto associativo e volontaristico, soprattutto nei territori di montagna e nei piccoli centri, davvero un grande problema. Conosco la sua sensibilità, signor Sottosegretario, perché l'ha dimostrata anche nei confronti dei nostri punti nascita; quindi sono certo che terrà conto di questa situazione, che va a favore della pratica sportiva e vorrei dire anche della sicurezza. Perché poi, se le società si sentono valorizzate e avvertono che la norma consenta loro di rispettarla, lo fanno; ma se sentono che la norma è troppo pericolosa, cercano di sfuggire alle responsabilità.

Signora Presidente, rispondo all'atto parlamentare del senatore Pagliari inerente alla situazione occupazionale della Simply SMA, società di proprietà della SMA SpA, facente parte del gruppo Auchan, con specifico riferimento ai punti vendita di Salsomaggiore Terme e Fidenza. Lo scorso 31 maggio, la Simply SMA ha comunicato ai 38 lavoratori interessati la chiusura dei punti vendita di Salsomaggiore Terme e Fidenza a far data dal prossimo 30 giugno. Le ragioni di tale scelta sono da ricondurre essenzialmente al fatto che negli ultimi anni i due punti vendita hanno registrato delle perdite significative con un *trend* sempre più negativo. La società ha altresì comunicato l'intenzione di provvedere alla ricollocazione dei 38 lavoratori presso alcuni punti vendita dell'*hinterland* milanese, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Nei giorni 6 e 20 giugno scorsi, presso la Provincia di Parma, si sono tenuti due incontri nell'ambito del tavolo interistituzionale - convocato dal Presidente della Provincia di Parma, nonché sindaco di Salsomaggiore e dal sindaco di Fidenza - avente ad oggetto la situazione dei 38 lavoratori dei punti vendita Simply SMA di Salsomaggiore Terme e di Fidenza. In tale sede, i vertici aziendali hanno rappresentato le ragioni che hanno determinato la decisione di chiudere i due punti vendita, mentre i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni locali hanno evidenziato lo scarso preavviso (un solo mese) con cui è stato notificato ai lavoratori il trasferimento in altri punti vendita (distanti fra i 110 e i 150 chilometri), con un sacrificio per alcuni impossibile da sostenere. Le rappresentanze sindacali ed istituzionali hanno, pertanto, richiesto un differimento di tre mesi della chiusura dei due punti vendita al fine di valutare la possibilità di accedere a strumenti di sostegno al reddito e di ricollocare i 38 lavoratori presso altri punti vendita presenti nella Provincia parmense, anche appartenenti ad altre catene commerciali. I vertici aziendali si sono riservati di valutare la richiesta. Informo, inoltre, che per la giornata di domani è prevista una nuova convocazione del tavolo interistituzionale al fine di pervenire di pervenire ad un accordo che, in conformità agli impegni presi dalle parti al termine del precedente incontro, possa definire le modalità per l'apertura di una procedura di mobilità, gli strumenti di sostegno al reddito applicabili e le misure volte alla ricollocazione dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali si sono riservate di sottoporre al voto dell'assemblea dei lavoratori il contenuto dell'eventuale accordo. In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza meramente locale della vicenda rappresentata con il presente atto parlamentare, posso comunque assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare la situazione e a seguirne l'evoluzione con la massima attenzione, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

di assistenza nella mobilità, perché la trattativa che sta andando avanti porterà probabilmente a uno slittamento del termine di chiusura, ma saranno poi necessarie misure a sostegno dei lavoratori, perché

mi preme evidenziare che il quadro normativo e regolamentare di riferimento per il settore della distribuzione di *gas* naturali risulta ad oggi completo degli elementi

da ultimo le linee guida richiamate nell'interrogazione medesima, e adottate con decreto ministeriale del 22 maggio 2014, hanno fornito le modalità operative da seguire nella determinazione del valore di rimborso spettante ai gestori uscenti all'atto dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio

ma non è ancora stata pubblicata la sentenza. A ogni modo, l'efficacia delle linee guida impugnate non è stata sospesa e alcune gare sono state avviate. Peraltro, proprio per tener conto di alcune difficoltà incontrate in questi primi avvii, è stata introdotta una ulteriore proroga ai termini ultimi per la pubblicazione dei bandi con decreto-legge del 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2016, n. 21. le difficoltà incontrate dagli enti locali e dalle stazioni appaltanti nella predisposizione e nel completamento dei bandi di gara sembrano essere causate non da un dato normativo regolamentare, ma piuttosto dalla determinazione del VIR in contraddittorio con i concessionari locali. Anche per ciò che attiene il quadro regolatorio predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica, il *gas* e il sistema idrico, esso risulta completo degli elementi necessari alla verifica dei dati tariffari, nonché alla formulazione del piano industriale da offrire in gara.

in discussione nelle Commissioni del Senato, i relatori, d'accordo con il Governo, hanno presentato un emendamento che prevede l'introduzione di alcuni meccanismi acceleratori del vaglio dei bandi e degli scostamenti VIR-RAB presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, laddove tali bandi risultano ovviamente coerenti con il quadro normativo e regolatorio vigente. Tale emendamento recepisce, tra l'altro, le indicazioni fornite congiuntamente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una recente segnalazione.

fondamentalmente rimaniamo insoddisfatti. È vero che alcuni bandi di gara sono finalmente pronti, ma il combinato disposto delle incertezze sulla valutazione dei rimborsi per gli impianti, dei tempi troppo stretti per risolvere i conflitti locali e dei contenziosi sulle linee guida continuerà a rendere le procedure di gara farraginose e a produrre ricorsi. Crediamo sia un caso che una delle prime gare indette - quella del Comune di Venezia - sia già stata sospesa dal TAR nello scorso maggio e analoghe difficoltà si prevedono per le gare di Comuni importanti come Torino, Milano, Varese, Roma, e altri. In sostanza, tutti gli elementi critici che avevamo sottolineato nella nostra interrogazione sono tutt'ora presenti e non se ne vede una soluzione. I ritardi che colpiranno la maggior parte delle gare, causati dai ricorsi, scarsa appetibilità dei ricavi tariffari, dei rimborsi e contenziosi vari, non faranno altro che creare danni alle società coinvolte e ai Comuni stessi. È mancata totalmente la capacità di governare con indicazioni chiare e scelte limpide questa fase di passaggio nell'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi. E chi ne fa le spese sono la libertà di concorrenza, i piani industriali di piccole e grandi imprese del settore, i lavoratori coinvolti che la sinistra continua a difendere a parole, ma a penalizzare nei fatti. Alla fine anche i cittadini ne fanno le spese. C'è un'altra valutazione da fare, seppure di massima: mancheranno tutti gli introiti che le nuove gare avrebbero dovuto portare ai Comuni e, quindi, i relativi investimenti sui servizi sui territori. Mancheranno le conseguenti tasse per lo Stato e, soprattutto, mancheranno tutte le plusvalenze

la nostra insoddisfazione, concludiamo sottolineando come, ancora una volta, ci troviamo di fronte a scelte sbagliate e contraddittorie che non vanno nella direzione di aiutare lo sviluppo e la competitività, ma che complicano e penalizzano la vita di imprese, Comuni e soprattutto i cittadini.

convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il Ministero dello sviluppo economico sta predisponendo il decreto per individuare le disposizioni per un processo un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. Le isole minori non interconnesse rappresentano una realtà particolare, caratterizzata da ecosistemi delicati e quindi protetti, grande variabilità della domanda di energia nel corso dell'anno, comunicazioni con la terraferma che in condizioni climatiche avverse possono essere difficili. La continuità del servizio è stata assicurata finora con una regolazione che riconosce le specificità delle isole, sia in termini di organizzazione della filiera (produzione, distribuzione, vendita), sia riguardo al riconoscimento dei maggiori costi della fornitura, mediante integrazioni tariffarie, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e poste a carico della generalità degli utenti elettrici. Date la specificità e la variabilità delle situazioni - come ho riferito - che si riscontrano nelle isole minori, si è ritenuto opportuno effettuare un apposito studio, affidato a Ricerca sul sistema energetico - RSE SpA, che fornisse elementi utili ad una migliore finalizzazione del decreto. Lo studio ha consentito di avere non solo un quadro adeguato riguardo alla struttura della produzione elettrica attuale, ma anche utili indicazioni sui consumi, sulle disponibilità di risorse rinnovabili locali, sugli scenari di diffusione delle fonti rinnovabili e sui relativi effetti economici. Inoltre, lo sviluppo tecnologico delle fonti rinnovabili e la conseguente riduzione dei costi rendono ora disponibili opzioni che, nei limiti possibili per garantire la sicurezza del sistema, possono assicurare la progressiva copertura della domanda con fonti rinnovabili, utilizzando, laddove necessario, la minore spesa conseguente alla riduzione della produzione tradizionale che - come detto - è sostenuta con specifiche integrazioni gravanti sulle bollette elettriche. Ciò premesso, entro pochi mesi dovrebbe essere completata la normativa di attuazione del citato decreto-legge n. 145 del 2013, che costituirà il quadro di riferimento per la promozione della copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse con il continente attraverso fonti rinnovabili. Riguardo al finanziamento della nuova centrale nell'isola di Favignana, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, non risulta alcun progetto finanziato a favore di SEA Favignana con il programma POI Energia. Relativamente al citato meccanismo di integrazione tariffaria applicato alle imprese elettriche operanti in alcune isole minori e al quale è soggetta anche la SEA Favignana SpA, evidenzio che il sistema prevede che la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), previa istruttoria sui dati di bilancio dell'impresa, reintegri in un determinato anno i maggiori costi sostenuti nell'anno precedente, come rilevati contabilmente nei bilanci d'esercizio (soggetti ovviamente a certificazione). Il meccanismo si fonda sull'esigenza, a parità di tariffa nel territorio nazionale, di ripianare gli extracosti di gestione sostenuti e non altrimenti recuperabili in realtà disagiate (nel caso, le isole minori non interconnesse caratterizzate da costi di produzione o gestione maggiormente rilevanti rispetto alla terraferma). la Cassa reintegra l'extracosto sostenuto sotto forma di integrazione tariffaria in favore delle imprese ammesse al regime, per consentirne il pareggio di bilancio e solo su dati di consuntivo (le erogazioni sono, per ragioni di continuità, a cadenza bimestrale con regolazioni di conguaglio annuali). Il meccanismo descritto non prevede forme di anticipazione e/o erogazione a fondo perduto a qualsiasi titolo, fatte salve eventuali esigenze specifiche individuate caso per caso e solo qualora disposte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) in qualità di regolatore e amministrazione vigilante di Cassa. Allo stato attuale la SEA Favignana ha ricevuto il conguaglio di integrazione tariffaria per l'anno 2012 e la Cassa per i servizi energetici e ambientali è in attesa dell'approvazione da parte dell'Autorità di di regolazione dell'aliquota per l'integrazione tariffaria a conguaglio per l'anno 2013. Posto che le regolazioni di conguaglio sono basate sui dati di bilancio del corrispondente anno, al momento si stanno coprendo a consuntivo i costi sostenuti fino al 2013, relativi quindi a periodi antecedenti alla attuazione di interventi di costruzione del nuovo impianto oggetto dell'interrogazione di cui si discute. Per le annualità successive la la SEA percepisce acconti bimestrali, basati sulle ultime aliquote definite secondo il meccanismo generale applicabile a tutte le imprese ammesse al regime di reintegrazione dei costi. Pertanto, non appare corretto affermare che la Cassa per i servizi energetici e ambientali abbia finanziato il progetto. Evidenzio che, qualora l'impresa abbia titoli autorizzativi (nel caso specifico di competenza della Provincia) - ferma restando l'esigenza da parte di Cassa per i servizi energetici di verificare l'allineamento dei costi di realizzazione ai costi di mercato e la congruenza dell'impianto con il contesto locale - la CSEA riconoscerebbe i costi di costruzione dello stesso impianto secondo i normali criteri di imputazione a bilancio. Il criterio guida è, infatti, l'esigenza di garantire la continuità e l'affidabilità della fornitura di energia elettrica sull'isola a condizioni analoghe al resto del territorio nazionale e a prezzi di fornitura unici nazionali. Infine, stante la vicinanza dell'isola alla terraferma, si è ritenuto opportuno un approfondimento sulle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, dell'interconnessione della rete elettrica dell'isola al sistema elettrico nazionale. A tal riguardo, è stata già effettuata una valutazione preliminare sulla fattibilità tecnica del collegamento elettrico e sui relativi costi. Si ritiene, tuttavia, necessario procedere a ulteriori approfondimenti, in particolare sugli aspetti economici dell'intervento in relazione ai potenziali benefici e sulle modalità operative più idonee alla realizzazione dell'interconnessione, anche tramite il coinvolgimento dei soggetti titolari del servizio di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica sul territorio della Sicilia. Da ultimo segnalo, senatore Santangelo, come da notizie apprese dalla direzione competente del Ministero

dice di no, ma probabilmente un finanziamento per altre vie arriva. Ciò premesso, si vuole costruire un'altra centrale per produrre 20 megawatt,